Signori senatori, è con sgomento vivissimo e con grande preoccupazione che abbiamo appreso dei gravissimi attentati avvenuti a Mumbai nella giornata di ieri. Accanto alla preoccupazione per questa nuova risorgenza di un terrorismo feroce che attacca indiscriminatamente vittime innocenti è forte il cordoglio per le numerose vittime di questi atti di barbarie. Un cordoglio che non possiamo non esprimere, in modo particolare, per l'efferato assassinio di Antonio de Lorenzo, nostro connazionale. Il presidente Schifani, a nome dell'Assemblea, ha già espresso tali sentimenti ai suoi familiari, insieme alla più ferma condanna per questo terrorismo crudele. Davanti a tragedie come queste possono sembrare inutili o rituali gli appelli alla tolleranza reciproca e alla pace. Questi appelli vanno, tuttavia, rinnovati uniti alla condanna più forte per un terrorismo che nessuna ideologia politica, religiosa o sociale può in alcun modo né giustificare, né comprendere. Così come tutti devono ribadire il dovere da parte della Comunità internazionale di impegnarsi fino a quando il terrorismo non venga definitivamente sconfitto. In segno di partecipazione al dolore dei familiari di Antonio de Lorenzo, ai quali va il nostro affetto e la nostra solidarietà, in ricordo della sua tragica fine e in segno di solidarietà verso tutte le vittime che ieri sono state colpite a Mumbai, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento.

***Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca***

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi... scusi, senatore Valditara. Prego i colleghi senatori di consentire al senatore Valditara di svolgere la relazione e a noi di ascoltarla;

Credo che una puntualizzazione importante debba essere fatta in occasione della trattazione di questo decreto-legge

dalla consapevolezza che l'università italiana non è il centro del malaffare. L'università italiana, nel bene e nel male, non si distingue da qualsiasi altro settore della vita pubblica italiana.

lo dicono prestigiose riviste scientifiche internazionali, lo dice un'indagine del Ministero dell'educazione nazionale francese, pubblicata su "Le Monde" nel febbraio 2007: internazionali, i ricercatori italiani vengono prima dei ricercatori francesi e tedeschi. Detto questo, sono innegabili tuttavia alcune criticità.

Detto questo, sono innegabili alcune criticità: una cattiva gestione delle risorse; sprechi di risorse, peraltro modeste; poca trasparenza; poca competizione; il problema della cosiddetta piramide rovesciata (40.000 professori a fronte di 20.000 ricercatori); un'ingessatura burocratica opprimente; la tendenza a trasformare le università italiane in superlicei dove si fa soprattutto didattica e pochissima ricerca e, devo aggiungere, un eccesso di spesa per un numero sempre più crescente di personale a fronte di una spesa del tutto inadeguata per le infrastrutture della ricerca.

Lanostra università - e il nostro sistema di istruzione in generale - è agli ultimi posti tra i Paesi più sviluppati per capacità di far sì che un ragazzo povero che entra nel sistema di istruzione possa uscire con le competenze per accedere alla classe media. È un sistema che configura una cristallizzazione sociale, un sistema che per molti aspetti è rimasto indietro negli anni. Molte delle riforme che oggi ci apprestiamo a varare sono già state affrontate dai principali Paesi europei dalla fine degli anni '90. In Italia, invece, sono state semplicemente abbozzate, in altri casi non sono mai state proposte.

Poi voglio anche aggiungere la legge 28 febbraio 1998, n. 31, sui concorsi, che è stata, a mio avviso in modo sbagliato, rieditata nel febbraio di quest'anno dal precedente Governo, che con i due idonei, idonei, il concorso locale e il membro interno certamente non favorisce quella richiesta di trasparenza che viene dalla società italiana. Voglio infine aggiungere che queste pratiche degenerative, sotto gli occhi di tutti, sono state, soprattutto la moltiplicazione irrazionale dei corsi di laurea, un portato del cosiddetto 3 più 2 che probabilmente andava pensato

(ben 150 corsi di laurea contano meno di 15 studenti), in tutto questo non è estranea la politica, che spesso e volentieri negli ultimi 15 anni ha difeso, sponsorizzato, sostenuto e talvolta persino imposto l'apertura di cattedrali nel deserto. Occorre dunque procedere ad un risanamento e ad un rilancio del settore. Ebbi a dire che il 2009 dovrà essere dedicato al risanamento e alle riforme strutturali importanti: dal 2010 occorrerà ragionare in termini di rilancio anche con riferimento alle risorse. Voglio anche sottolineare che è mancata, a partire dall'inizio degli anni Novanta, una grande visione culturale. Negli ultimi 15-20 anni molte delle riforme sono state troppo spesso effettuate sotto la spinta dell'emergenza, senza un quadro strategico ed è giusto invece avere ben presenti alcuni forti criteri di riferimento.

all'interno di un sistema fondato sulla competizione tra atenei che abbia due grandi finalità: la promozione sociale degli studenti attraverso una formazione adeguata e la contribuzione allo sviluppo di una innovazione del sistema produttivo. Da qui è partito il Governo, da qui siamo partiti con questo decreto-legge. E voglio entrare subito nel vivo della trattazione. Quando abbiamo detto «applichiamo finalmente una legge dello Stato», la cosiddetta legge Berlinguer del 1997, che prevedeva l'obbligo di non superare il 90 per cento nel rapporto tra spese per il personale e fondo di finanziamento ordinario, abbiamo fatto cosa attesa dalla parte sana del mondo universitario e da essa richiesta, perché in nessun Paese al mondo si spende quasi esclusivamente per stipendi e quasi nulla per ricerca e infrastrutture di ricerca.

delle facoltà mediche, probabilmente la stragrande maggioranza delle università italiane avrebbe un rapporto pari al 100 per cento o molto

le risorse vengono impiegate soltanto per pagare stipendi, l'università è costretta ad indebitarsi o a chiedere soldi ai privati o ad aumentare le tasse universitarie. È quindi evidente che chi fosse contrario ad una misura di questo tipo si assumerebbe la responsabilità di dire «aumentiamo le tasse», «privatizziamo l'università italiana», «indebitiamo l'università italiana». Il provvedimento in esame contiene anche una marcata apertura ai giovani. Innanzitutto, voglio ricordare un punto che nel dibattito politico è quasi scomparso, ma che credo sia particolarmente importante: come dicemmo già dall'inizio della legislatura, occorreva sbloccare le assunzioni per 2.800 ricercatori che sono in attesa di entrare nel mondo della ricerca.

che credo rappresenti un obbligo morale cui anche l'attuale opposizione nella passata legislatura aveva cercato, senza riuscirci, di

che chi è di condizioni modeste non debba andare a lavorare per potersi mantenere nell'università. Voglio sottolineare che lo stanziamento previsto dal Governo in questo decreto è doppio rispetto a quanto non sia stato stanziato negli ultimi anni,

che applica una misura di questo tipo. Le risorse devono andare soprattutto a quelle università che per qualità della ricerca e della didattica sviluppino risultati positivi. risultati positivi. Nella scorsa legislatura avevamo già presentato, con numerosi colleghi che siedono in Parlamento, proposte emendative in questa direzione. Sono altrettanto compiaciuto che la Commissione abbia approvato oggi l'introduzione dell'anagrafe delle pubblicazioni scientifiche che consente di certificare con grande chiarezza le pubblicazioni di professori e ricercatori, di avere un quadro chiaro. Sono particolarmente soddisfatto per il fatto che si introduce una autentica rivoluzione che d'ora in poi gli scatti automatici di stipendio non verranno più liquidati automaticamente, ma saranno condizionati alla pubblicazione scientifica nell'ultimo biennio. Sono anche soddisfatto perché nelle Commissioni giudicatrici entrerà soltanto chi negli ultimi anni ha effettuato pubblicazioni scientifiche. È assurdo che un professore possa giudicare altri senza aver mai pubblicato nulla. Credo che questa sia una iniziativa fondamentale per dare concretezza e serietà. Sono inoltre particolarmente soddisfatto che le università ed i rettori, in sede di bilancio consuntivo, abbiano l'obbligo di dire con grande trasparenza

Si introduce quindi il meccanismo del sorteggio. Non credo nell'effetto taumaturgico del sorteggio. Credo, invece, che il sorteggio abbinato all'elezione possa essere un segno di moralizzazione efficace. È un segnale e, in quanto tale, senz'altro positivo. Ovviamente la vera riforma dovrà essere fatta in un confronto ampio con il mondo universitario, con l'opposizione; a mio avviso, una riforma dovrà necessariamente passare da una lista di idonei a numero chiuso, entro cui sviluppare una chiamata diretta.

il rilancio del dottorato ed anche - consentitemi di aggiungere - i contratti individuali sul modello tedesco, anche qui sviluppando quello che oggi già facciamo in questo decreto, pagando di più i professori che lo meritano. Voglio evidenziare un ultimo aspetto: il mondo universitario nelle audizioni si è espresso in modo favorevole sul decreto. Voglio ricordare le parole del presidente della CRUI Decleva, del presidente Lenzi, le aperture importanti del presidente Morcellini,

un settore interessato ad una riforma anche pesante, che comporterà dei costi per qualcuno, per qualcuno, dà il suo sostanziale appoggio. Credo che sia un segnale molto importante. Mi auguro che anche altri settori della vita pubblica italiana sappiano fare altrettanto, come sta facendo la parte più consapevole e rappresentativa dell'università italiana che sta collaborando ad un rilancio del nostro sistema e a far sì che finalmente anche il nostro mondo universitario possa essere al pari degli altri sistemi più avanzati e che possa contribuire a creare sviluppo, benessere e crescita complessiva per il nostro Paese. colleghi, intervengo per palesare tutta la contrarietà del mio Gruppo parlamentare al provvedimento in questione. Il Gruppo Italia dei Valori infatti non può che essere contrario oltre che nel merito anche, e non di poco conto, nel metodo utilizzato anche questa volta, per arrivare a fissare delle norme per degli importanti settori della nostra società. L'aggettivo "urgenti" ricorre da mezzo secolo nel titolo dei provvedimenti legislativi che riguardano l'università. A parte la necessità tecnica legata alla decretazione governativa, non è difficile riconoscere nell'impiego ricorrente della parola una sostanziale miopia nell'affrontare i problemi dell'alta formazione nel nostro Paese. Infatti, nel metodo, la maggior parte dei provvedimenti di cui si parla riguardano quasi esclusivamente il corpo docente e nel merito rivelano la cronica carenza della volontà politica di risolvere lo spinoso tema del precariato. infatti partire da lontano, quando l'estensione dell'accesso all'università a tutti i diplomati di scuola media superiore di durata quinquennale (1969) fu fronteggiata attraverso il ricorso spregiudicato agli incarichi di insegnamento. Lo Stato non intendeva sostenere in modo strutturale il costo della liberalizzazione. Nel successivo decennio 1980-'90 il DPR n. 382 del 1980, tentò di affrontare i nodi della situazione universitaria, anche con importanti innovazioni riguardanti la docenza come l'introduzione del ruolo dei professori associati (seconda fascia docente), la riapertura dei concorsi liberi a scadenza biennale per ordinari ed associati, con programmazione nazionale, e l'istituzione dei ricercatori, con limitata funzione docente dopo la conferma in ruolo. Il DPR n. 382 del 1980 segnò certamente una svolta nella trasformazione dell'università italiana in strumento democratico di promozione sociale, senza pregiudizio della sua fondamentale vocazione culturale. Tuttavia, parte per insufficiente valutazione delle difficoltà operative, parte per eccessiva fiducia nelle capacità di autoriforma del corpo accademico, lasciò irrisolti molti problemi, compresa la definizione dello stato giuridico dei ricercatori e la dinamica tra la domanda e l'offerta di alta formazione. Nel 1989 veniva emanata la direttiva europea che consentiva il riconoscimento, sul piano professionale, in tutti i Paesi membri della CEE, dei titoli di studio conseguiti dopo un corso universitario di durata triennale. I provvedimenti adottati dal legislatore alla fine degli anni '80 risposero all'orientamento europeo con l'istituzione dei corsi di diploma universitario triennale (DU) e la modifica della struttura della docenza, consistente nell'estendere anche ai ricercatori confermati

Infatti, dopo alcuni tentativi falliti nella XII legislatura, veniva consentito l'affidamento per contratto di tutti i corsi di insegnamento (1998). Veniva al pettine, negli stessi anni, la necessità di rivedere il meccanismo dei concorsi

attribuiti direttamente agli atenei, con l'ulteriore potere di designare un membro delle commissioni. Ancora una volta il legislatore puntava la propria attenzione sul reclutamento dei docenti delle fasce superiori, mentre continuava a lasciare insoluto il problema dello stato giuridico dei ricercatori, trovando anche modo, in uno degli ultimi articoli della legge, di rendere ufficiale «*una* *limitata* *attività* *didattica*» La legge n. 230 del 2005 riprendeva ed aggiornava lo strumento della programmazione degli atenei, legandovi anche le richieste di nuovi posti di docenza, con commissioni giudicatrici formate con sistema misto

con i suoi tagli alle risorse ordinarie e l'inedito e sconcertante avvio dell'abdicazione da parte dello Stato all'alta formazione dei cittadini. La parte finanziaria del provvedimento infatti configura un intervento doveroso ma estemporaneo. la necessità e l'urgenza di intervenire al fine di assicurare la distribuzione di risorse, a partire dall'anno accademico in corso, attraverso disposizioni che rendono selettivi i finanziamenti destinati ai concorsi già banditi, oltre quelli che si bandiranno, ai sensi delle nuove nonne, entro il 30 novembre, nonché la necessità ed urgenza di intervenire - nelle more di un riordino dei criteri di reclutamento dei professori universitari - sulle procedure concorsuali e sull'esclusione degli enti di ricerca, "erroneamente inclusi", o non esplicitamente esclusi, dal in tutta sincerità è inaccettabile che si decida di normare questo settore in questo modo! Con questo contenuto e con ulteriori tagli e, quando non ci sono quest'ultimi, ovvero quando son previste nuove risorse, esse sono coperte in modo non corretto,

che avranno raggiunto meglio specificabili obbiettivi. Allo stesso modo, il Gruppo Italia dei Valori non può essere completamente felice, pur registrando certamente una inversione di tendenza, rispetto alla previsione contenuta all'articolo 3 del provvedimento. Il mio

Il decreto-legge n. 180 non sembra presentare le caratteristiche di necessità e di urgenza previste dalla Costituzione, ma è piuttosto volto ad intervenire per rimediare parzialmente ad alcuni errori tecnici, presenti nella legge n. 133, senza peraltro intaccare minimamente i tagli finanziari. Si tratta dunque di un provvedimento minimale il cui aspetto migliore, rispetto al taglio di un miliardo e mezzo di euro previsto dalla legge n. 133, è stata l'attesa, l'annuncio, la comunicazione che si sarebbero date risposte serie alle università italiane. Ma, come nel leopardiano «Il sabato del villaggio», «la speme e la gioia» lasciano presto il posto al «travaglio usato». In realtà è talmente palese il livello minimale di questo decreto - com'è stato detto con parole chiare dal collega professor Veronesi nel dibattito in Commissione che, rispetto ad emendamenti necessari, votati all'unanimità dalla 7a Commissione per evitare centinaia di ricorsi scontati, questa mattina la Commissione bilancio ha preteso di aggiungere ovunque l'espressione chiarissima «senza alcun onere aggiuntivo». legge n. 133, con i suoi tagli di un miliardo e mezzo di euro, domina e sovrasta questo provvedimento e possiamo affermare con chiarezza che «la montagna ha partorito il topolino».

È un primo provvedimento di apertura che però, se non sostenuto da altre iniziative che modifichino i tagli dei trasferimenti del 46 per cento nel 2010, sarà irrilevante».

perché il 2010, cui ha fatto riferimento anche il relatore, è dietro le porte, anzi, è già nella programmazione delle università. In questo autunno 2008 ci si potrebbe chiedere se l'università italiana ha anche un futuro. Tra i Paesi europei dell'OCSE, infatti, l'Italia è ultima per investimenti nell'università, sia rispetto al PIL, che rispetto alla spesa pubblica nazionale. Il sistema universitario attraversa, inoltre, una profonda crisi di credibilità, sotto attacco da parte dei mezzi di comunicazione. E vorremmo che fosse causale il fatto che in soli tre giorni, su proposta del presidente Quagliariello, che peraltro non fa parte della 7a Commissione, su iniziativa del presidente Possa e su decisione del presidente Schifani, sia stata autorizzata una Commissione d'indagine relativa ai bilanci e agli sprechi delle università: strana un'indagine conoscitiva che presuppone già un risultato ed un obiettivo che sembrano finalizzati immediatamente a questo decreto e ai tagli della legge n. 133 . Lo diciamo perché questo, con molto amor di Patria per il nostro Parlamento e per il nostro Governo - e dico nostro! - non serve all'immagine dell'Italia e dell'università italiana all'estero, non serve alla nostra credibilità all'estero, né a diminuire la tensione verso quelle famiglie, quegli studenti, quei docenti e quei rettori che chiedono risposte serie alla politica italiana. La terapia del Governo è chiara: ridurre ulteriormente e drasticamente sia i finanziamenti statali che il personale, e spingere gli atenei ad un'autoprivatizzazione, con l'illusione che «il cavallo affamato e privatizzato» ricominci a galoppare.

dunque, la natura pubblica del sistema universitario, ed ho detto pubblica, non statale. Il ruolo dello Stato, come erogatore e garante di un sistema di alta formazione, è indispensabile per assicurare le condizioni affinché l'università resti e divenga sempre di più elemento centrale dello sviluppo del Paese e del suo stesso *welfare*.

rispondere che noi non abbiamo paura del reclutamento, ma ci siamo solo accorti che questo provvedimento era fatto così male (e per questo motivo è stato modificato in Commissione)

interrogasse un altro professore in portoghese: ci sembra proprio una scelta logica, pensata bene e in maniera razionale. Noi non abbiamo paura di un sorteggio che, così limitato, rischia di provare gli stessi vizi già sperimentati con il ministro Fontana a metà anni Ottanta.

che non ha una grande preparazione si saprebbe chi lo ha assunto o chi ha suggerito la sua assunzione. Quindi, nessuno ha paura. La senatrice Garavaglia e l'onorevole Veltroni proporranno un nostro disegno di legge sul reclutamento. Gli articoli 2 e 3 sono indubbiamente positivi ma, casualmente, limitati solo al 2009 senza un piano triennale.

vi sono interventi utili: il numero ed il tempo a nostra disposizione in Commissione - quasi uguale a quello usato dalla maggioranza - testimoniano che il relatore, se è arrivato in Aula, lo è per scelta nostra, del Partito Democratico, dell'Italia dei Valori e di tutta l'opposizione,

Parlando, circa un anno fa, ai responsabili di scuola e università del partito, Gian Felice Rocca, vice presidente per l'*education* di Confindustria, disse a tutti (di centro-destra e di centro-sinistra) che un Paese che taglia finanziamenti alla scuola, all'università e alla ricerca fa bassa manutenzione e non investimento. Ecco le parole giuste, che riprendo per il provvedimento in esame: è una bassa, ordinaria manutenzione, non un investimento in speranza.

una presa di coscienza, un segnale, un'immediata ed urgente prospettazione di un'inversione di tendenza. Credo che questo lo abbiano riconosciuto anche i colleghi dell'opposizione, risparmiandoci, in quest'occasione, il consueto rito democratico - civilissimo, per carità - delle pregiudiziali di costituzionalità.

di baroni, baroncini e baronastri che cosa fu? Il massimo dei profili di irresponsabilità. La piramide rovesciata è una tragedia, non soltanto per il numero dei professori rispetto a quello dei ricercatori, ma per il fatto che due intere generazioni sono state pregiudizialmente escluse dall'accesso alla ricerca scientifica per tutelare e garantire meglio magari quelli della mia generazione. Voglio dire questo perché un giornale, nei giorni scorsi, annunciava che nell'Aula del Senato si sarebbe rivista rivista in opera la congiura dei baroni; non credo sia così: mi fido del relatore

Quando, nel 1968, un ministro bravo e riformatore, l'onorevole Gui, presentò il

pur di non accettare l'incompatibilità Parlamento-cattedra, civettavano con il docente unico. E nei datzebao, quando avevo vent'anni, c'era scritto «Viva la lunga lotta del popolo vietnamita» (io ero per gli Americani), «del popolo palestinese» (io ero per Israele), «dei braccianti e dei metalmeccanici» (io ero per Croce e non per Gramsci), e «degli assistenti universitari»! Ecco la saldatura tra lo squadrismo dei baronastri e la congiura dei baroni: mi auguro che in questa occasione, né quest'Aula, né le condizioni del Paese, consentano più quella tragedia. Per riscuotere quella tragedia, senatrice Garavaglia, bisogna ora aspettare la generosa impostazione del pianista Pedini e la realizzazione di un antico uomo di scuola, Salvatore Valitutti,

degli ordinari di portoghese che non sono sufficienti, ma certo abbiamo acquisito troppi portoghesi dell'ordinariato. Vi sono dei profili di irresponsabilità rispetto ai quali il relatore,

- e certamente il professor Giavazzi ha tutto il diritto di chiedere sul «Corriere della Sera» un provvedimento di emergenza - ma questo provvedimento, che si vota come agenda Gelmini, con tutto il rispetto che si

Signor Presidente, devo dire che ai toni da Masaniello dell'amico Compagna ho preferito assai i toni misurati, anche se

Ricordo che la nostra università nell'ultimo decennio ha aumentato le immatricolazioni nonostante un declino del numero dei giovani tra i 18 ei 20 anni. La nostra università ha più che raddoppiato il numero dei laureati. Erano 140.000 nel 2000 mentre oggi sono 300.000. La loro qualità è qualità è peggiorata? Non sappiamo perché non esistono analisi in questo senso. Non lo si può dire, ma certamente la produttività dell'università è notevolmente migliorata.

Bisogna certamente rimediare agli sprechi, alla divisione, molto netta, tra università di qualità mediocre e università di qualità eccellente; bisogna agire nel profondo.

sistema concorsuale, eliminando la doppia idoneità - che avrebbe semplificato enormemente le cose - piuttosto che congegnare un marchingegno che certamente non funzionerà e creerà moltissimi problemi. come è stato proposto in Commissione - un'estrazione secca dei candidati giudici delle commissioni. Anche questo avrebbe semplificato enormemente le procedure.

Credo che qui qualcuno osi finalmente accostare le parole "università" e "merito", dopo molti anni in cui l'autonomia senza responsabilità - come è stato ricordato - ha generato troppi docenti e burocrati, costi di funzionamento, scarse risorse per la ricerca ed, infine, anche alti costi per gli studenti. Gli applausi vengono da chi, come me e come tanti colleghi, ha lavorato per molti anni nell'università in Italia ed all'estero; vengono da tutti i colori che non ne possono più di vedere il duro lavoro e i buoni risultati di molti, ed in particolare di tanti validi giovani che attendono meritate opportunità di accesso, vanificati da norme che introducono e diffondono il malcostume, con concorsi pilotati dove non solo si sa prima chi vince, ma si sa prima anche che chi vince è spesso un cretino. Poi ci stupiamo se si arriva al sesso offerto in cambio di esami da parte di studentesse e studenti, che evidentemente imparano che con questi metodi si può fare strada nella vita.

Va avanti chi merita nell'assegnazione delle risorse: le università meno efficienti sono punite (il criterio del 90 per cento potrà non essere perfetto, ma in qualche modo si doveva pur cominciare!);

che mai come in questo caso sarebbe l'emblema di una resistenza dei vecchi interessi corporativi. Le commissioni saranno composte da soli ordinari, principalmente sorteggiati anziché eletti. Vi saranno si escluderanno associati e ricercatori che sono ricattabili nelle commissione - bisogna dirlo! - recidendo l'assurdo groviglio che oggi permette ad un candidato in un concorso "x" di sedere contemporaneamente ai suoi stessi giudici nella commissione di un concorso

luogo, un decreto, al di là da venire ma imminente, stabilirà nel dettaglio i parametri internazionali con cui saranno valutati per titoli e pubblicazioni i candidati ricercatori. Tali parametri sono noti ed applicati da anni in tutto il mondo: se saranno introdotti sul serio in Italia, non solo innalzeranno la qualità del reclutamento, ma daranno speranze speranze e certezze a chi si impegna, produce ottime pubblicazioni ed oggi è alla mercé di commissioni combinate, capaci di preferire candidati mediocri, dalle qualità spesso inconfessabili. Infine, va avanti chi merita

e facendo fino ad oggi dell'università, al contrario di quanto dovrebbe essere in un Paese civile, un ostacolo all'uguaglianza delle opportunità e una grave fardello per la crescita culturale, civile ed economica del Paese.

Il fatto positivo è che il Governo, dopo i primi atti su scuola ed università, si è dovuto fermare e ha dovuto prendere atto della forte opposizione nel Parlamento e nel Paese ai provvedimenti che riguardano tutto il sistema sapere. Il Governo ha dovuto ascoltare, anche se lo ha fatto solo in minima parte e dando risposte davvero frettolose, talmente frettolose che molti colleghi della maggioranza sono intervenuti in Commissione a denunciarle, come abbiamo fatto noi, su molti punti. Il Governo ha dovuto prendere atto che un *turnover* al 20 per cento, come previsto dal decreto-legge n. 112, avrebbe comportato un blocco delle carriere e del reclutamento e sarebbe stato troppo penalizzante per i giovani, per i ricercatori e per i docenti: certamente il 50 per cento è più ragionevole. Il Governo, ancora, ha dovuto prendere atto che esiste un problema del diritto allo studio in questo Paese, che esiste un problema di pari opportunità e di uguale cittadinanza e che resta ancora inattuato il dettato costituzionale che prevede che tutti i meritevoli possano accedere all'alta formazione. all'alta formazione. Voglio ribadire un concetto emerso nella discussione che abbiamo svolto in Commissione. Se il nostro Paese vuole dare un minimo contributo alla costruzione della società della conoscenza, cui ci chiama l'Europa, e valorizzare i talenti dovunque si trovino, indipendentemente dalla provenienza sociale, deve investire sul diritto allo studio e promuovere la mobilità sociale che, praticamente, oggi è inesistente nel nostro Paese.

Ma, certo non possiamo perdere di vista il contesto generale in cui si collocano questi provvedimenti.

il primo, abbiamo potuto osservare - anche qui oggi ne abbiamo avuto qualche dimostrazione - che una buona parte della maggioranza descrive l'università con un'immagine tutta negativa, un'università fatta tutta di baroni, di baronie, di nepotismo, di corruzione. Ci è venuto il sospetto che si tratti di un'immagine costruita ad arte in maniera da giustificare i tagli eccezionali operati dal Governo, provvedimenti depressivi, punitivi, come ha detto poco fa il senatore Livi Bacci; l'università va punita. Ebbene, noi non la pensiamo così! Detto questo, non vogliamo neanche affermare che nell'università va tutto bene. Assolutamente no. Bisogna riconoscere criticità che esistono e che vanno corrette per recuperare appieno il senso della missione dell'università, missione dell'università, che consiste nell'alta formazione, nella ricerca migliore più avanzata possibile, nel contribuire alla competitività del Paese. Se questa è la missione, però, non si può neanche mettere tutto nello stesso calderone e dire che nessuna di queste funzioni viene svolta dalle nostre università, dai nostri ricercatori, dai nostri docenti universitari soltanto per arrivare a giustificare i tagli. Di questo infatti

studenti e ciò è dimostrato dal successo che i nostri laureati riscuotono all'estero. I nostri ricercatori sono tra i più produttivi in Europa;

mondo. Nelle nostre proposte rovesciamo la prospettiva, partiamo dal dare valore alle eccellenze per meglio correggere le criticità e far prevalere il merito, per far prevalere la produzione scientifica, la valutazione, l'offerta didattica, la preparazione dei nostri studenti. Tutti sanno che esiste un problema di valutazione seria e di premialità delle università che producono di più e meglio, però però la definizione di università virtuose non può riferirsi prevalentemente o esclusivamente allo sfondamento o al non o al non sfondamento del tetto del 90 per cento dell'utilizzo dei fondi per il personale, trascurando proprio la produzione scientifica. Ma proprio questo si fa nell'articolo 1 del decreto-legge escludendo, in base a questi criteri, da una parte dei fondi e dal reclutamento, le università cosiddette non virtuose. Vengo alla seconda dimensione di quel contesto di cui parlavo prima, ossia i tagli gravissimi

in pratica quelle premialità che pure sono previste per le più virtuose, perché tutte le università saranno in difficoltà e nessuna di loro potrà essere virtuosa in base a quei criteri. Sono previsti - lo voglio ricordare, perché sembra che sia scomparso dall'orizzonte della nostra discussione - 700 milioni in meno nel 2010 e 800 milioni in meno nel 2011. Se non si corregge questo dato, è inutile parlare di qualsiasi riforma. C'è il rischio che norme così severe penalizzino a tal punto le università da rendere difficile per loro realizzare anche i piani di rientro già previsti per quelle che hanno sfondato quel famoso tetto del 90 per cento; nessuna di loro riuscirà mai più a ridiventare o a diventare virtuosa. C'è il rischio che ottime università, eccellenti università del nostro Paese si impoveriscano anche sul piano della produzione scientifica e questa credo che debba essere la nostra maggiore preoccupazione in questo momento.

di sopprimere il comma 4 dell'articolo 1 che si occupa di questo problema e presentare, da parte del Governo o dei colleghi della maggioranza (lo stesso faremo noi ovviamente), un disegno di legge sul reclutamento da discutere in maniera approfondita, con la speranza e con la possibilità di arrivare ad una proposta condivisa. Credo che nessun sistema di reclutamento sia buono in assoluto; abbiamo sperimentato negli anni scorsi diverse combinazioni fra elezioni e sorteggio, eppure siamo ancora qui a discuterne. Il problema è che dobbiamo davvero inventarci, creare e arrivare a regole certe, basate sulla premialità e sulla sanzione, che arrivino quasi a costringere a reclutare i migliori e non quelli che sono magari più vicini al maestro sia sul piano della

nei concorsi sono previsti due idonei e non un solo vincitore, come noi avevamo chiesto di fare, per esempio, l'anno e purtroppo poi invece il Parlamento ha cambiato questa misura. Allora perché non prevedere nel provvedimento il vincitore unico dei concorsi? Penso che in questo modo si contribuirebbe davvero a introdurre una nuova dimensione di una nuova etica pubblica che farebbe bene anche alle università. *(Applausi dal

sottolineato in tutti gli interventi dell'opposizione - si vuole dare una qualche giustificazione ai tagli che sono stati inclusi nella finanziaria, ma non sono assolutamente provvedimenti necessari a fare tutto quello che, invece, è emerso dagli interventi dei rappresentanti della maggioranza, a cominciare dal relatore. Infatti, la madre di tutte le battaglie, se si vuole parlare di riforma invece che di mero aggiustamento di decisioni relative a quella che oggi - ahinoi - continua ad essere chiamata *governance*, che è qualcosa che attiene al dominio dell'amministrazione e non al dominio retorico della politica (che è ben altra cosa, cioè prendere delle decisioni radicali di vera e propria riforma), è l'abolizione del valore legale dei titoli di studio. Senza questo tutto il resto, la mancanza di responsabilità o il controllo della spesa sono vana coloritura spesa sono vana coloritura di misure totalmente inesistenti e sicuramente inefficaci dal punto di vista del cambiamento nel nostro sistema universitario. Sono convinto che il senatore Compagna si riferisse alla prima guerra di Indocina, quando lui aveva vent'anni e leggeva i datzebao; allora si fece lo sbaglio di non prendere in considerazione, da parte americana, un Ho Chi Minh che diceva «aiutatemi» in chiave antisovietica e si preferì allearsi con un antidemocratico per sconfiggere i comunisti. Ebbene, oggi si rischia di fare la stessa cosa; non si prende in considerazione ciò che invece è fondamentale: includere all'interno dell'università italiana la libertà.

È stato portato l'esempio della mancanza di docenti di portoghese per tenere concorsi relativamente a questa materia e si è detto che non si possono mandare insegnanti di spagnolo a effettuare questo tipo di selezioni. Ricordo che siamo uno dei 27 membri dell'Unione europea: perché non prendere in considerazione la possibilità di rivolgersi al Portogallo per far arrivare professori che sicuramente meglio di altri possano valutare la qualità della competenza linguistica di chi in quella materia dovrà ottenere il dottorato o una cattedra?

solo attraverso una partecipazione ampia all'interno del contestodell'Unione europea possiamo non soltanto arricchirci dell'esperienza degli altri Paesi,

- che sarà purtroppo, credo, emendato molto poco nel prosieguo del nostro dibattito - è totalmente contrario, proprio perché si continua a volare basso, volare basso, e volando basso non si fa l'interesse di nessuno. Ho sentito parlare anche di misure per il rientro in Italia dei cosiddetti cervelli che sono stati costretti a fuggire: bene, spero che quando si parlerà di una riforma più organica di questa - che però non può non partire dall'abolizione del valore legale dei titoli di studio - si ascoltino questi cervelli e si faccia capire ai nostri cervelli (e ce ne sono in Italia) quali sono le condizioni che questi avrebbero studiando o lavorando all'estero e quali invece sono quelle che si vanno ad offrire a coloro che si verrebbero far rientrare in Italia a 1.800 euro al mese.

Signora Presidente, Ministro, Sottosegretario, onorevoli senatori, la Lega Nord non è mai stata e mai sarà a favore dei baroni universitari che, negli ultimi anni, hanno utilizzato le facoltà per assumere gli amici degli amici non curandosi di potenziare il profilo professionale dei docenti e di elevare la qualità della ricerca italiana ed inducendo i veri cervelli, magari figli di non potenti, ad emigrare all'estero. Con questo intendo affermare che la Lega Nord non ha alcun conflitto d'interesse e pertanto noi possiamo porci quali garanti dell'effettiva concretizzazione dello spirito e degli obiettivi che il decreto in discussione vuole perseguire, ponendoci in una prospettiva di ampia collaborazione con tutte le forze politiche che vogliono assicurare la creazione di un'università meritocratica, trasparente, efficiente e vicina agli interessi degli studenti. La conversione in legge del decreto-legge n. 180 vuole introdurre il principio di responsabilità delle singole università rispetto alla gestione dei fondi e rispetto al mantenimento degli equilibri di bilancio in ottemperanza al principio dell'autonomia responsabile di ciascun ateneo. Introduce misure di controllo del *turnover*, atte a ribaltare la cosiddetta piramide rovesciata che oggi vede l'università italiana gravata da un numero elevato di professori ordinari contro un numero non adeguato di ricercatori, per lo più precarizzati, con gravi pregiudizi per i risultati della ricerca. Introduce il meccanismo del sorteggio per la composizione delle commissioni di valutazione per il reclutamento di professori e ricercatori, introducendo elementi di trasparenza nel passaggio chiave del reclutamento stesso. Ciò indica il chiaro messaggio che si vuole limitare il proliferare di fenomeni di clientelismo, familismo, inefficienza e spreco che, penalizzando l'università italiana, in più gravano sul bilancio dell'intero Paese. Fissare criteri oggettivi e trasparenti per la valutazione significa migliorare la gestione delle risorse dello Stato e dotare il sistema di più efficienza. Oggi le commissioni di concorso per il reclutamento dei docenti universitari e dei ricercatori sono composte solo per elezione da parte di docenti e ricercatori di pari grado. Il meccanismo dell'elezione rende possibili accordi e scambi di voti che permettono la composizione controllata delle commissioni. Inoltre la valutazione dei candidati è a discrezione dei commissari, non esiste nemmeno una graduatoria finale dei partecipanti e l'accesso agli atti è consentito solo previo avvio di un'azione legale. Introduce, inoltre, misure di monitoraggio della qualità del sistema universitario, vincolando l'erogazione dei finanziamenti a criteri di effettiva incidenza verso le esigenze della società ponendo al centro lo studente. Il decreto-legge n. 180, infine, fissa elementi di meritocrazia per facilitare il diritto allo studio e l'accesso all'università per gli studenti più capaci e meritevoli. Sia pure in un contesto economico complessivo che suscita preoccupazioni e che rischia di pesare anche sugli sviluppi dell'università nei prossimi anni, tali aspetti introducono elementi di rottura rispetto alle logiche corporative, familistiche e di sperpero di risorse pubbliche che hanno ispirato tante scelte negli ultimi decenni. La Lega Nord vigilerà proprio sul mantenimento dell'integrità di questi aspetti anche in sede di elaborazione dei regolamenti e della prossima riforma universitaria. Noi non vogliamo che prevalgano bizantinismi tecnici, così come non accettiamo le proteste ispirate a motivazioni ideologiche e a volontà disfattista, volte unicamente a mantenere lo *status quo*. Mi limito a citare la presa di posizione del Consiglio universitario nazionale che, al di là dei proclami di facciata a sostegno del decreto-legge n. 180, nella mozione del 19 novembre boccia l'introduzione del meccanismo del sorteggio per la formazione delle commissioni per il reclutamento di professori e ricercatori, auspica il ripristino della composizione delle commissioni antecedente n. 180 e che le assunzioni dei ricercatori a tempo determinato siano sottratte a qualsiasi forma di regolamentazione ministeriale. La Lega Nord ha in serbo per il Ministro tante altre richieste e proposte a favore degli studenti universitari, per una università italiana che possa confrontarsi con quella internazionale senza arrossire perché al passo con le direttive europee e con gli standard raggiunti dagli altri Paesi dell'Unione europea e per un utilizzo efficiente e razionale delle risorse economiche ed umane. Esse saranno esplicitate con chiarezza e determinazione nel momento in cui sì procederà ad una vera ed articolata riforma universitaria, che il ministro Gelmini si è impegnata a presentare nel prossimo futuro. Nel frattempo, il decreto-legge n. 180 deve essere ritenuto un primo valido passaggio volto a sbloccare i concorsi di assunzione che ormai si rendevano urgenti, purché non venga stravolto nella sua connotazione innovativa. Per questo la Lega Nord si appella al senso di responsabilità morale di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, rispetto ad un settore così determinante per lo sviluppo del Paese. *(Applausi

ancora una volta stiamo esaminando un provvedimento d'urgenza, un decreto-legge, invece di un provvedimento più ragionato. Si toccano alcuni punti di una materia complessa, quella della politica scolastica ed educativa,

le varie università fra loro. È una riforma a costo zero ma, stranamente, non viene mai messa in atto. Nell'attuale situazione bloccata dell'università ogni meccanismo che si vorrà mettere in atto, sia per la selezione di nuovi ricercatori sia per la progressione di carriera, temo possa risultare inutile e illusorio: si cambia tutto per non cambiare nulla. Le singole università dovrebbero invece poter avere autonomia reale e totale. Ogni università, con finanziamenti pubblici e privati, dovrebbe essere autonoma e stabilire criteri propri per la selezione dei ricercatori e dei professori, venendo pesantemente penalizzata in caso di comportamenti abolire i concorsi, abbandonare le logiche del pubblico impiego, con più contratti a tempo determinato (anche per cinque anni) che a tempo indeterminato. I progetti di ricerca da finanziare dovrebbero essere poi valutati da un'agenzia della ricerca che vagli l'attività scientifica dei ricercatori proponenti attraverso un sistema di *peer* *review* a livello internazionale, con un controllo rigido dei conflitti di interesse. Sappiamo di vivere un periodo di crisi, non del mercato ma nel mercato: operare dei tagli in questi momenti può essere anche un utile spunto per apportare innovazione e quei cambiamenti radicali di cui parlavo all'inizio dell'intervento per andare alla radice di un sistema malato. Sono momenti di grave difficoltà che spesso fanno sì che sia l'esterno a costringere ad un cambiamento. Ecco perché invito a valutare l'opportunità di elaborare strategie per attrarre capitali privati, italiani e stranieri, per il potenziamento dei nostri atenei, anche attraverso agevolazioni fiscali per coloro che investono nell'università e nella ricerca. In Italia i finanziamenti pubblici per la ricerca scientifica sono inferiori alla media OCSE, ancor meno sono gli investimenti privati; per questo è necessario andare oltre la mentalità secondo cui solo lo Stato può gestire l'università e la ricerca. Senza investimenti privati il nostro Paese rimarrà sempre un nano a livello internazionale: i soldi pubblici, in assenza di competitività, non basteranno mai e continueranno ad essere più volte sprecati.

*(PD)*. Signora Ministro, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, stiamo discutendo di un provvedimento che,

suppone ed evoca argomenti di grandissimo rilievo, se è vero che siamo nel secolo dei saperi, nella società della conoscenza; se è vero che attorno al tema delle culture si giocherà non solo un orpello, un *maquillage*, del nostro presente o del nostro futuro, bensì il cuore stesso della società che stiamo immaginando, globale e locale insieme. Di fronte allo spirito di Lisbona, alle medie dell'OCSE, e più in generale alla spinta che in tanti Paesi oggi non casualmente si ha e si pone verso gli strumenti formativi, noi stiamo procedendo,

va letto in controluce. Esso non sarebbe immaginabile, ma neppure chiaro alla lettura, se non vi fosse il fantasma di quella legge n. 133, che studenti e insegnanti, donne e uomini di varie generazioni, hanno messo in discussione con piattaforme alternative, tutt'altro che

immaginari significativi per un futuro che è soprattutto quello delle generazioni più giovani.

strutturazione delle nuove figure sociali, ma scatta la spinta, per così dire, baronale, quella dei concorsi; sì, è molto trasversale. Vorrei Vorrei anche aggiungere che mi ha colpito una certa polemica, un po' faziosa, su temi che hanno, invece, contraddistinto, semmai, chi ha per tanti anni governato questo Paese e anche quel Governo Berlusconi che

dalla parte più bassa della piramide, perché per andare in alto dobbiamo avere tanti bravi ricercatrici e ricercatori, che oggi sono largamente precari, quando va bene,

su questo o quel segmento del sapere, difficilmente l'autore è un consolidato professore ordinario, senza nulla togliere, ci mancherebbe; spesso è un giovane ricercatore che,

spesso con il presidente Possa - questa suddivisione metodica oggi sia forse anchilosata e degna di essere superata. Per quanto riguarda il diritto allo studio, non si può parlare spavaldamente di aumento indistinto delle sedi universitarie, piuttosto che dei corsi.

alle sedi universitarie come veri e propri luoghi attrattivi delle coscienze delle generazioni più giovani (o anche meno giovani, visto che la vita oggi giustamente si allunga),

Quante sono, invece, le spese che si potrebbero spostare, le risorse che potrebbero essere investite più utilmente per la formazione e la conoscenza! in una situazione in cui sempre di più la conoscenza e i saperi sono merci particolarissime e delicatissime, e non sono semplicemente un accumulo cognitivo, bensì anche - questo è il grande tema ed il rischio della modernità e postmodernità - nuovi strumenti strumenti di gerarchizzazione e segmentazione sociale. Quando si corre il rischio che all'antica contraddizione tra chi ha e chi non ha se ne aggiunga una, ancor più virulenta, tra chi si sa e chi non sa, si può creare una miscela esplosiva, drammatica, tragica. E qui non c'entrano la destra o la sinistra: c'entra un Paese che ha voglia di guardare al mondo con animo non marginale o con quello di una vecchia "Italietta",

per mettere qualche tappo ad una diga che non regge. Siamo innovatori: vorremmo più cultura, più conoscenza e più investimenti in questa enorme novità

infatti, è l'istituzione più alta per la cultura di un Paese, per costruire, con lo sviluppo civile, anche lo sviluppo economico.

perché tocca a questa nostra istituzione, Ministro, salvare le altre. Senatrice Aderenti, non può esserci conflitto di interessi se siamo qui a lavorare e a legiferare per il Paese.

secco potrebbe inserire tra gli esaminatori persone che, per tanti motivi, non hanno raggiunto gli stessi livelli degli esaminandi. Soprattutto, non si è tolta la seconda idoneità, che rappresenta lo scandalo della trattativa. Per un un candidato che vince il concorso ve n'è un altro già pronto per essere chiamato in un'altra università. Vi rendete conto di come è stata spiegata male all'opinione pubblica questa vicenda? Vi rendete conto che non è un sistema migliore degli altri e non possiamo accettarlo a lungo? Sono sicura che il Governo metterà mano ad un disegno di legge organico, nel

chiede attenzione a tutti sul merito, sugli strumenti di valutazione e sulla meritocrazia. Un decreto come questo, signor Ministro, allora sarebbe stato davvero ben servito se fosse stato urgentemente attivato l'ANVUR in servizio, altrimenti anche la distribuzione dei finanziamenti,

onorevoli colleghi, ringrazio la Presidenza per avermi dato la parola in questi cinque minuti, nonostante non avessi previsto né chiesto di intervenire in discussione generale. Ma, dopo la relazione eccellente e non reticente del collega Valditara, che condivido totalmente, e dopo aver ascoltato il dibattito, ho chiesto di intervenire perché francamente, le ipocrisie ultradecennali della sinistra italiana dentro l'università non possono adesso concedere spazio a interventi da mammole che vengono ad indicare i presunti rimedi taumaturgici dell'università italiana. Parlo ovviamente nella veste di senatore della Repubblica, ma prevalentemente nella veste di barone universitario per 38 anni nell'università italiana

come genitore - se permettete - di giovani ricercatori italiani che da anni lavorano brillantemente all'estero per affermare la propria professionalità e la propria autonomia mentale, intellettuale e di ricerca, che non è consentita nelle università italiane ad oggi. Vorrei affrontare

il passaggio dei concorsi dal livello nazionale a quello locale, per il vecchio sistema, nel quale - almeno - i vincitori corrispondevano al numero dei posti, contro il nuovo sistema che dava tre idonei. E dicemmo E dicemmo - oltre 15 anni fa, dopo la riforma Ruberti - che avremmo distrutto e bloccato l'università italiana per i vent'anni successivi, impedendo ai giovani ricercatori italiani di lavorare decentemente nel nostro Paese, ovviamente con il risultato

(il vincitore e un idoneo) avrò il 90 per cento di probabilità, nella mia disciplina, di dirle chi vince il concorso e chi sarà l'idoneo. senza ipocrisie, proprio perché chi parla ha avuto per tanti anni il ruolo di barone e ha combattuto perdendo sempre queste battaglie. Sto dicendo che la mia personale esperienza è una battaglia contro la sinistra italiana e il sindacato, che hanno voluto occupare l'università in questo modo. Questa è la realtà storica. È un problema italiano creato dalla sinistra italiana. mi permette di dare una testimonianza personale all'Aula? Questa è la mia versione, vissuta quotidianamente all'interno di ben quattro sedi universitarie: Torino, Milano, Bologna e "La Sapienza" di Roma.

titolo di merito per l'acquisizione dei finanziamenti. Questi ultimi in questi vent'anni sono stati distribuiti nel seguente modo: arrivano alle facoltà e ai dipartimenti tot milioni (allora di lire, oggi immagino di euro)

noti editorialisti su noti quotidiani nazionali: forse non tutti sanno che quei noti editorialisti pontificano sull'Italia, su qualunque cosa, essendo titolari di cattedra presso la Harvard University. Sono tutti amici, francamente, ma questa è la realtà. In conclusione, signora ministro Gelmini, lei ha fronteggiato con grande fermezza e coraggio questo argomento, un argomento che negli ultimi quarant'anni ha fatto cadere diversi Governi della Repubblica perché sono prevalse le commistioni, fino all'ultima, l'autonomia, che ha portato all'assurdità di considerare la laurea

che sono anche professori, ma non si sa se frequentano o meno le aule universitarie, che sostengono che l'università è ormai allo sfacelo. Non ci sto. Non ci possiamo stare.

Ministro, che l'università non è al capolinea per un motivo molto semplice. Come si fa a spiegare che all'estero i nostri studenti sono ricercatissimi? Le parlo da padre anch'io. Anch'io ho una figlia a New York da tre anni;

con cui ha condotto il dibattito sia in Aula, che in Commissione e per la disponibilità ad un confronto pacato e serio dimostrata. Credo che con questo provvedimento abbiamo inaugurato un metodo che, voglio sperare, potrà ripetersi anche nel futuro.

Signora Ministro, devo dare atto al Governo che ha rovesciato tutte le peggiori invettive che abbiamo ascoltato in queste settimane. Non è vero, dunque, che per il 2009 ci saranno tagli:

i nuovi fondi per il diritto allo studio e per le residenze, la deroga al blocco delle assunzioni per i 2.800 ricercatori, la deroga al blocco delle assunzioni per gli enti di ricerca, l'incremento dal 20 al 50 per

che si prosegua oltre con questo metodo che non è certo coerente con un criterio di efficienza e di uso corretto dei soldi pubblici. È stato detto, inoltre, che

un edificio e, ovviamente, dovrà pagare delle rate di mutuo che, però, sono inferiori rispetto all'affitto che per quello stesso edificio il Politecnico pagava. Ebbene, secondo il criterio che qualcuno di voi ha esposto dovremmo penalizzare il Politecnico perché ha ha operato una scelta virtuosa. Certamente si è indebitato, ma questo è un indebitamento positivo nel rapporto spese per il personale-fondo di finanziamento, abbiamo un parametro del 65 per cento, il che vuol dire che il Politecnico di Milano usa il 35 per cento delle risorse per svolgere ricerca per finanziare la possibilità concreta per gli studenti, per esempio, di accedere a delle biblioteca di eccellenza. Credo che anche da questo punto di vista sia necessario evitare qualsiasi confusione. aggiungere un'ultima questione che penso sia assolutamente indispensabile sottolineare. Il meccanismo della valutazione è fondamentale proprio per iniziare ad invertire quella tendenza per cui i soldi venivano distribuiti a pioggia, perché oggi sappiamo perfettamente che il criterio principale di distribuzione delle risorse è quello del numero di studenti iscritti in una determinata università. Questo non è un criterio meritocratico.

Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, un settimanale da sempre piuttosto severo con il nostro Paese e con la maggioranza che oggi lo guida, «The Economist», all'indomani della presentazione del decreto-legge in esame, ne ha parlato in maniera lusinghiera. Lo ha definito, dopo aver descritto in maniera impietosa il nostro sistema universitario, come un serio tentativo di cambiamento, insomma come una buona notizia per gli studenti e per quei docenti che interpretano l'insegnamento accademico e la ricerca come una missione determinante per il Paese. Spero che il Parlamento voglia confermare questa buona notizia e darne altre e di migliori, a partire dall'approvazione degli importanti emendamenti, assolutamente condivisi dal Governo, sottoscritti dal senatore Valditara, che ringrazio in qualità di relatore, unitamente al presidente Guido Possa e a tutta la Commissione, per la sua opera scrupolosa e attenta e per la ferma volontà di guardare ai mali del sistema per correggerli. Mi auguro che questo sia il primo passo verso la rivoluzione di un sistema che oggi appare, ed è, Spero nell'aiuto del Parlamento, di una maggioranza salda nella spinta riformatrice e di una opposizione da cui sono arrivate utili ed apprezzate indicazioni in sede di Commissione e, mi pare di poter dire, una generale comprensione dello spirito di fondo che anima il decreto, affinché ogni ateneo possa dare un contributo di qualità al futuro dell'Italia. Affrontiamo questo dibattito sotto gli occhi attenti del Paese, di un'opinione pubblica frastornata dalle inchieste che hanno messo sotto accusa alcuni esempi di cattiva gestione e di involuzione del sistema universitario. Oggi, con questa legge possiamo dare all'Italia il segno di una svolta, all'insegna del rigore e del riconoscimento del merito. Dobbiamo farlo per il futuro di tutti noi, noi, ma soprattutto per dare giustizia alle migliaia di validissimi studiosi che insegnano e fanno ricerca nei nostri atenei, e che non meritano certo di essere accomunati in una censura, talora in ogni caso sopra le righe, che riguarda solo un malcostume circoscritto. Sono e resto convinta che l'università italiana abbia bisogno di meno regole e comunque di regole che liberino le energie dei suoi migliori talenti, in primo luogo dei giovani. Come ebbe a ricordarmi la senatrice Finocchiaro nel corso del precedente dibattito, citando il Vangelo di Giovanni, "all'inizio era la parola". Oggi le parole di questo decreto costituiscono l'inizio di un cambiamento più volte tentato e sempre rimasto incompiuto; e mi piace qui ricordare tra i miei predecessori il ministro Ruberti, autore allora contestatissimo delle norme sull'autonomia universitaria, il ministro Berlinguer e il ministro Moratti, i cui tentativi di coniugare a quell'autonomia l'inscindibile concetto di responsabilità e il riconoscimento del merito costituiscono il filo di continuità con gli interventi che intendo promuovere; una continuità che rivendico, che ho inteso rappresentare, nella scorsa legislatura, presentando un ampio disegno di legge sul merito; una continuità che fa da sfondo alle linee guida appena presentate, cui abbiamo intenzione di legare i provvedimenti in questa legislatura. Non mi illudo che non ci siano proteste. Ci sono corporazioni che reagiscono all'attacco ai loro interessi consolidati e cercano di opporsi, a partire da questo decreto, ad ogni ipotesi di reale cambiamento. Ebbene, col vostro aiuto, queste corporazioni non vinceranno. Oggi noi iniziamo a curare alcune piaghe di quel sistema. Iniziamo a curare, in maniera non definitiva ma certamente salutare, viste le reazioni che gli articoli del decreto hanno provocato, la piaga di prassi concorsuali giudicate universalmente inidonee a selezionare i migliori docenti, impedendo che sia un sistema inadeguato ad immettere in ruolo alcune migliaia di docenti. Sono consapevole del fatto che il sistema del sorteggio presenta limiti e problemi, non maggiori né minori di tutti i complicati sistemi concorsuali che sono stati provati in Italia negli ultimi decenni. In questo momento, l'esigenza prevalente era però quella di dare un netto segnale di discontinuità rispetto ad una prassi ormai insostenibile, ma di farlo limitando al massimo il disagio e i ritardi per le migliaia di studiosi che del tutto legittimamente attendono da tempo di partecipare ai concorsi, bloccati ormai da tre anni per una decisione del precedente Governo. Mi rivolgo al ministro-ombra Garavaglia, per dire che mi sarebbe piaciuto poter eliminare la doppia idoneità, ma in questo caso sono stata fortemente dissuasa dall'ufficio legislativo, che ha portato solide motivazioni di un rischio concreto di ricorsi che avrebbero portato al blocco dei concorsi. È solo per questo motivo che all'interno del decreto non è stata eliminata la stortura della doppia idoneità. Il metodo che abbiamo adottato rappresenta quindi una misura di emergenza strettamente *una tantum* e insieme l'ennesima dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno, che un sistema universitario ampio, complesso e multiforme non può più reclutare i docenti con strumenti che risalgono ad epoche molto lontane e molto diverse. Come indicato nelle linee guida, intendo aprire immediatamente un confronto ad ampio raggio con il mondo accademico e il Parlamento per riflettere con spirito profondamente riformatore su come voltare pagina. Mi auguro che questa sia davvero l'ultima volta in cui il Governo, il Parlamento e le università sono costretti a dibattere su alchimie concorsuali lontane anni luce dalle esigenze di una università libera e moderna e di un Paese che da essa si attende un esempio e un modello. Iniziamo a dire che autonomia non significa, non può più significare arbitrio nella gestione dei fondi per il funzionamento degli atenei, perché dobbiamo esercitare lo stesso rigore che ogni amministratore pubblico ha il dovere di esercitare quando gestisce il denaro della collettività. Iniziamo a porre il merito, soprattutto quello misurato dalla qualità della ricerca scientifica, come criterio per la ripartizione di una quota significativa dei fondi statali, cento già nel 2009, una quota che vogliamo far diventare sempre maggiore, sino al 30 per cento, invertendo un *trend* che ha privilegiato esclusivamente la spesa storica. Iniziamo a dire basta se, come mi auguro, verranno approvati alcuni emendamenti, a un meccanismo di automatismi di anzianità slegato dalla produzione scientifica. Iniziamo a riaprire le porte dell'università ai giovani e a riequilibrare un corpo docente, che negli ultimi anni sembra aver pensato soprattutto alle esigenze di chi già era all'interno del sistema rispetto a quelle dei giovani meritevoli che aspiravano ad entrarvi. A questi cambiamenti il Governo crede davvero: per questo ha incrementato in modo cospicuo le risorse che gli atenei potranno impiegare già a partire dal 2009 per nuove assunzioni, soprattutto per quelle di giovani ricercatori. Ora dobbiamo fare uno sforzo collettivo per dimostrare che la volontà di riforma del sistema universitario è convinta e radicata: è in questo modo che potremo impostare su basi nuove le discussioni sui finanziamenti statali a partire dal 2010. Ci sono nel decreto numerose altre novità di rilievo: ne segnalo solo due. Diamo maggiori certezze ai ricercatori degli enti pubblici, perché pure in mezzo al rigore economico

l'*iter* per le chiamate dirette dall'estero, eliminando ogni tetto numerico, ed estendendole anche agli enti di ricerca. L'obiettivo non è tanto quello di far rientrare gli studiosi italiani, ma, più ambiziosamente, quello di far sì che tutti gli studiosi possano considerare l'Italia una sede accogliente per condurre le loro ricerche: dobbiamo ritornare ad essere a pieno titolo una delle capitali del sapere nel mondo, aperta ai migliori talenti. Ma nell'onda della protesta ci sono i giovani, che pure del sistema che vogliamo abbattere sono vittime, cui è stato raccontato che il cambiamento è l'opposto di quello che in realtà è. Io ho sotto gli occhi le loro proteste, ma più ancora il loro futuro. Accolgo anche le loro critiche più aspre perché sono convinta di seguire le leggi del giusto. Ma a loro dico di non cadere nel grande inganno, di non confondere il diritto allo studio col diritto a conseguire un pezzo di carta, che è invece lo svilimento dello studio. Noi vogliamo dire basta ai pezzi di carta, basta a strumenti utili, forse, solo per partecipare a qualche concorso pubblico. Noi vogliamo che la laurea torni ad essere la dimostrazione di una fatica compiuta, la prova di una cultura e di una capacità conseguita. Noi diciamo sì al precetto costituzionale che ci chiede di garantire ai meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei più alti gradi dell'istruzione. Non solo 65 milioni di euro ci consentiranno di finanziare ulteriori progetti per residenze universitarie, ma 135 milioni di euro in più per il fondo di finanziamento delle borse di studio consentiranno (se le Regioni faranno, e ne sono certa, il loro dovere) di dare quanto la Repubblica deve loro a tutti gli aventi diritto, a tutti gli studenti meritevoli e privi di mezzi. Onorevoli senatori, si tratta in questo senso dell'incremento di risorse più forte di sempre. L'ultimo incremento significativo su quel fondo avvenne 3 anni orsono ad opera del ministro Moratti, ed era stato di 30 milioni. Oggi molti, troppi, di coloro che hanno diritto alla borsa di studio non la ricevono. Ancor più vergognoso è che questa situazione sia a macchia di leopardo. Mentre in Lombardia, Piemonte e in altre (poche) regioni tutti gli studenti idonei ricevono la borsa di studio, in media, più del 20 per cento idonei non riceve la borsa di studio per mancanza di fondi; ed in alcune regioni del Meridione, proprio dove ce ne sarebbe più bisogno, questa percentuale di ingiustizia supera il 50 Questo articolo del decreto mi sembra la migliore risposta a chi, in buona o in mala fede, ha dichiarato che la legge n. 133 tagliava i fondi per il diritto allo studio. Così non era. E il decreto di cui vi chiedo l'approvazione fissa un indirizzo esattamente opposto a quanto propagandato. Onorevoli senatori, il Paese ci chiede, in tutti i campi del nostro agire politico, rigore, serietà, utilizzo oculato delle risorse, segnali forti di un cambiamento da rendere irreversibile. Mi auguro, e sono convinta, che noi tutti vorremo essere all'altezza di queste aspettative.

del presidente onorario di Fondiaria SAI, Salvatore Ligresti, e gli assessori comunali di Firenze, Graziano Cioni e Gianni Biagi,

Per chi non lo sa (forse anche questo Governo si tappa oltre che le orecchie anche gli occhi), l'imprenditore Ligresti è uno dei soci CAI che è stato già condannato a due anni e tre mesi di detenzione. Ripeto, è da sempre che chiediamo con forza di

di nuovo indagato per ipotesi di corruzione e questa persona dovrebbe essere uno degli esponenti del rilancio di tale compagnia. Ecco perché, signora Presidente, mi rivolgo e continuo a rivolgermi al Capo dello Stato, perché qui c'è una sordità assoluta sia del Governo che del Parlamento.

da ambiti degni di fede che il giudice fallimentare del tribunale di Roma competente per il fallimento dell'Alitalia avrà come consulente lo studio del dottor Fantozzi, già commissario straordinario della stessa Fonti certe informano inoltre che lo stesso Fantozzi percepirà la cifra di 16 milioni di euro per il suo incarico come commissario straordinario; di tale notizia si sta già interessando la trasmissione

sulla rassegna stampa di ieri (e non ce l'ho con la rassegna stampa ma con il tipo di informazioni che essa dà) non si è parlato del fatto che il capo della segreteria di Matteoli, un ministro della Repubblica, è stato indagato per un reato gravissimo, quello di

Presidente, senatori, sono stata informata poco fa che a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, città nella quale vivo, è crollata la facciata di un vecchio edificio in ristrutturazione, compresa l'impalcatura su cui lavoravano due dipendenti dell'impresa edile. I due operai non sono attualmente in pericolo di vita, certo è che ancora una volta il lavoro è diventato pericoloso e che certamente occorre più attenzione all'applicazione delle norme delle leggi in materia di sicurezza. La Protezione civile è intervenuta nell'immediato evacuando anche l'edificio scolastico adiacente, dimostrando un grandissima professionalità, insieme alle autorità sanitarie. Ci auguriamo che non si aggiungano altri feriti nella prossima ora. Il Gruppo dei senatori della Lega Nord è vicino ai feriti ed alle loro famiglie e chiede al Governo di accertarsi che abbiano un'adeguata assistenza sanitaria, e non solo. La Lega Nord chiede alla magistratura di fare chiarezza al più presto sull'incidente, individuando le responsabilità. **Per

credo si possa rimanere ostaggi del disinteresse sulla materia di un Gruppo e quindi non si arrivi alla formazione di questa Commissione. Potrebbe essere serio, visto che qui si parla di meritocrazia e di trasparenza, fissare una data entro la quale chi non ha fatto il nome dei commissari non parteciperà alla Commissione.

ha parlato dello scandalo che sta travolgendo l'amministrazione comunale di Firenze, il cui sindaco Dominici è anche Presidente dell'associazione nazionale dei Comuni italiani. è che il senatore Pedica - non so in base a quale ragionamento - ha per sfortuna del senatore Pedica, io sono anche consigliere comunale di Firenze tale vorrei dire al collega di documentarsi un po' meglio, perché l'indagine della magistratura riguarda comportamenti degli assessori del comune di Firenze.

per informare il senatore Pedica - una commissione comunale di inchiesta e abbiamo chiesto di sospendere l'approvazione del piano strutturale, che doveva essere approvato a giorni. Proprio oggi, inoltre, abbiamo chiesto le dimissioni del sindaco e quindi il commissariamento del Comune di Firenze. Il Governo, caro esponente dell'Italia dei Valori, non c'entra proprio niente.